"La Stampa") - su politici e tecnici amici. Si parla di soldi e nella bufera sono finiti Aldo Cosentino, direttore generale del Ministero dell'ambiente ed Emilio Brogi, attuale capo della segreteria del ministro Matteoli. Per i magistrati dell'antimafia calabrese

Signor Presidente, ho l'impressione che l'opposizione voglia continuare sul piano dello scandalismo e utilizzare notizie giornalistiche

scandalistiche, provocatorie, utilizzando strumenti antichi che conosciamo perfettamente, non possano trovare spazio all'interno di quest'Aula.

agroalimentare***